Il testo del disegno di legge n. 1720 è stato già esaminato e approvato, articolo per articolo, dalla 8a Commissione permanente in sede redigente. Il relatore, senatore Cicolani, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

una breve relazione evidenziando alcuni contenuti necessari per spiegare ai colleghi e all'opinione pubblica alcune questioni che in queste settimane sono apparse più volte sulla stampa. prima di tutto sui tempi complessivi di questo provvedimento e sul modo con cui abbiamo lavorato nonché sulla scelta

Abbiamo ricevuto il testo di questo provvedimento di riforma di alcuni articoli del codice della strada dalla Camera,

immaginando che il Governo successivamente sarebbe intervenuto con un'ampia revisione dello stesso. Abbiamo quindi ereditato questo testo circa nove mesi fa, alla fine del mese di luglio dello scorso anno. Tenendo conto dei periodi feriali e delle elezioni regionali, che complessivamente hanno impedito per circa tre mesi l'esame di questo provvedimento, nonché della sessione di bilancio, che a sua volta ha impedito per circa due mesi di esaminare il provvedimento, l'8a Commissione ha lavorato su questo disegno di legge per circa quattro mesi. In questo periodo sono state svolte oltre 45 audizioni e, a valle di queste, i colleghi senatori hanno presentato circa 400 tra emendamenti ed ordini del giorno: mai, nessun emendamento con una volontà ostruzionistica, tutti costruttivamente elaborati per concorrere al miglioramento del codice. È stato proprio questo immenso lavoro che ha determinato il Governo e la Commissione a non limitare l'esame soltanto ai punti punti affrontati nella discussione presso la Camera dei deputati, ma a cogliere anche l'occasione per una completa revisione del codice della strada, pur sapendo che sarebbe stato un lavoro molto importante ed oneroso per la Commissione. Di questo oggi trattiamo: portiamo all'esame dell'Aula un complessivo riesame del codice, che è derivato dall'ascolto di un enorme numero di attori e da una stretta collaborazione tra Commissione e Governo sull'esame di ogni singolo emendamento. Per dare un'idea dei 400 tra emendamenti ed ordini del giorno presentati oltre 100 sono stati approvati: questo vuol dire che il contributo

completamente la discussione in Aula avrebbe sicuramente portato ad una dilazione ulteriore dei tempi e all'impossibilità di arrivare ad una definizione della revisione del codice della strada prima dell'esodo estivo.

a me spetta rivolgere un ringraziamento particolare a tutti Gruppi della Commissione per la qualità, oltre che per la quantità, del lavoro svolto. Sottoponiamo quindi all'Aula queste novità del codice.

alla possibilità che i veicoli eccezionali siano accompagnati da personale di tipo ausiliario e non da personale della Polstrada. Abbiamo

altresì introdotto la necessità del certificato storico delle patologie del richiedente. Per le patenti professionali abbiamo introdotto l'obbligo dei test di alcol e droga anche nel caso di revisione della patente. Siamo intervenuti - cosa tentata varie volte in quest'Aula - sui proventi delle sanzioni per alta velocità,

Questi proventi, che sono evidentemente aggiuntivi per lo Stato rispetto a quelli che attualmente vengono incassati, e l'insieme dell'inasprimento delle sanzioni che pure produciamo attraverso questo provvedimento, come di avere delle risorse che vengono destinate in parte al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per incrementare le dotazioni per la manutenzione

Abbiamo inasprito le sanzioni per gli autotrasportatori che violano i tempi di riposo, anche quando eccedono quote minimali dei tempi di guida; su questo c'è stato, quindi, un inasprimento sanzionatorio che ha escluso le lievi sforature dei tempi di guida. Abbiamo introdotto l'obbligo di indossare il casco per i conducenti di biciclette per i ragazzi fino a quattordici anni. Abbiamo anche introdotto la possibilità di accedere, pur se soltanto per una volta, ai lavori di pubblica utilità in sostituzione di pene detentive e pecuniarie per chi ha guidato sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, ma senza mai provocare incidenti. Abbiamo anche stabilito il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle stazioni di servizio autostradali. autostradali. Questo divieto, come potete leggere dal testo, mentre per le bevande superalcoliche è generale, per le bevande alcoliche è limitato alle ore notturne.

di convergere verso un unico codice della strada europeo. A questo fine l'agenzia sarebbe uno strumento indispensabile, secondo noi. Non potendo istituirla, al di fuori di questo contesto, abbiamo istituito perlomeno un comitato di coordinamento presso il Ministero che tenga conto dell'attuazione delle norme del codice della strada e delle problematiche che ne scaturiscono, considerando il fatto che la gran parte delle strade oggi è in mano alle Regioni e agli enti locali. Ciò al fine di fare una politica comune, coordinata e raccordata con questi enti sia sulla segnaletica, sia sulla normazione generale del traffico all'interno di tutto il territorio nazionale.

abbiamo facilitato l'acquisto e l'utilizzo degli apparecchi di controllo remoto da parte degli enti locali; abbiamo introdotto la targa personale e una serie di norme che combattono le intestazioni fittizie delle auto

per chi trasporta un animale ferito di derogare ad alcune norme del codice - anche se ciò verrà regolato da un apposito decreto ministeriale - al fine di soccorrerlo, con la la possibilità di dimostrare anche successivamente questa circostanza. Abbiamo introdotto, ed è un fatto molto rilevante, anche se

Abbiamo eliminato la norma che toglieva i punti dalla patente per le infrazioni compiute in bicicletta e abbiamo introdotto nuove norme in ordine alle competizioni sportive,

previo un allungamento della sospensione della patente (quindi non si tratta di una diminuzione della pena), di concedere delle ore, fino a un massimo di tre al giorno, per ottemperare a questa finalità.

fatto. A valle di questo lavoro, abbiamo prodotto circa 25 elementi di novità ed abbiamo approvato anche ordini del giorno importanti,

a molte associazioni - in particolare l'Associazione italiana familiari e vittime della strada - che chiedono paletti più stretti per i giudici in ordine alle circostanze aggravanti e attenuanti,

il provvedimento al nostro esame, in materia di sicurezza stradale, arriva nell'Aula del Senato dopo un lungo ed impegnativo lavoro svolto nella Commissione lavori pubblici,

abbiamo ascoltato, proposto, ragionato, corretto e ricorretto il testo, lavorando senza anteporre le ragioni partitiche al buonsenso, almeno nella maggior parte dei casi. In alcuni articoli è emersa un'evidente diversità di impostazione, dovuta ad una diversa visione delle problematiche e delle loro ricadute sociali, che potremmo anche chiamare semplicemente "diversità culturali". tratta di quella diversità politica che delinea, prima di ogni altra valutazione nel merito, il campo del centrosinistra dal campo del centrodestra. Malgrado questo e malgrado il fatto che su diversi articoli avremmo voluto un altro tipo di definizione, possiamo dire che il testo uscito dalla Commissione migliora l'attuale codice della strada e migliora, a nostro parere, anche il testo che ci è giunto dalla Camera dei deputati, rendendolo più aderente alle necessità dei nostri concittadini. Proprio per queste ragioni riteniamo che il tempo impiegato per lo svolgimento delle numerose audizioni e per la discussione di tutte le proposte emendative al testo sia stato un tempo speso bene. Riassumendo, per dare un giudizio politico del lavoro svolto in sede redigente, il Partito Democratico ha scelto di proporre una sua relazione di minoranza non tanto per distinguersi, ma per informare l'Assemblea e i cittadini di quanto è stato condiviso con convinzione, di quanto è stato proposto dal Partito Democratico e poi accolto e di quanto invece ci vede in posizione critica.

il testo, tra gli aspetti maggiormente positivi del provvedimento si segnala, in via del tutto sommaria, l'accoglimento di diverse proposte presentate dal Gruppo del PD che, sin dall'avvio dell'esame degli emendamenti, erano state dichiarate prioritarie. Tra queste si ricorda innanzi tutto il lavoro di pubblica utilità, cioè l'introduzione di pene alternative alla pena detentiva e alle pene pecuniarie per la guida in stato di ubriachezza o a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti. Spesso chi è sottoposto a procedimento penale con questi titoli di reato non sconta mai la pena o la sconta dopo sette-otto anni, quando diventa definitiva. Con questa norma il giudice, addirittura con decreto penale di condanna, può proporre all'imputato di svolgere i lavori di pubblica utilità per tutto il tempo previsto dalla pena detentiva, che altrimenti - ripeto - non verrà mai Naturalmente, il beneficio viene riconosciuto solo a chi non ha causato con il proprio comportamento un incidente stradale, e può essere concesso una sola volta. Praticamente, con la revoca del provvedimento di confisca dell'auto facilitiamo un percorso immediato di riabilitazione. Ovviamente, nel caso in cui il giudice procedente dovesse valutare che gli obblighi di lavoro di pubblica utilità vengono violati, dispone il ripristino immediato della pena detentiva. Inoltre, si introduce l'obbligo per gli esercizi pubblici (e in via prioritaria per i locali di intrattenimento

per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test prima di mettersi alla guida; sono previsti altresì idonei spazi di riposo. l'inasprimento delle sanzioni per chi utilizza i ciclomotori e le minicar con motore modificato; il divieto di utilizzo delle minicar per i soggetti cui è stata ritirata la patente, la patente, l'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza per chiunque guidi una minicar. Vi è poi la previsione finalizzata a far sì che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità con l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni siano attribuiti per cento all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e per il restante 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore. Nella versione originaria del testo pervenuto dalla Camera dei deputati i proventi erano ad esclusivo appannaggio dell'ente proprietario della strada, con ciò arrecando pregiudizio non solo ai bilanci dei Comuni, ma soprattutto sul livello e l'intensità dei controlli sulla nostra rete stradale. Ancora, in tema di educazione e buone pratiche di guida, si segnala la previsione dell'obbligo di dare comunque la precedenza ai pedoni quando questi si accingono ad attraversare le strisce pedonali: questa norma sicuramente in parte l'indirizzo risarcitorio. Da ultimo, vorrei segnalare l'approvazione di un ordine del giorno con il quale il Governo è stato impegnato ad istituire anche nel nostro Paese, come è già avvenuto in gran parte dei Paesi comunitari, un'apposita Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, alla quale verrà assegnato il compito di garantire una maggiore tutela degli utenti della rete stradale nazionale ed una più efficace attività di sviluppo, manutenzione e gestione della medesima, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dettati dalle norme comunitarie. Numerose altre misure apportano un complessivo miglioramento del nostro codice della strada, che in più parti viene aggiornato alle esigenze emergenti nella nostra società. Tuttavia, malgrado i numerosi aspetti positivi introdotti, il giudizio sul provvedimento rimane condizionato da talune scelte adottate dal Governo, contrastanti con il clima positivo maturato in Commissione lavori pubblici, in particolare su alcune specifiche tematiche rispetto alle quali vi era un comune giudizio positivo. Tra queste si lamenta, in primo luogo, il mancato accoglimento delle proposte direttamente mirate ad accrescere il livello dei controlli necessari a garantire una maggiore sicurezza stradale. In particolare, dopo una lunga discussione in Commissione, il Governo ha posto il veto sull'approvazione di un emendamento finalizzato a garantire la piena funzionalità dei vari organi di polizia stradale con specifico riguardo alle attività di intensificazione dei controlli stradali, la repressione dei comportamenti e delle infrazioni alla guida, nonché il controllo sull'efficienza dei veicoli. Sono note le difficoltà della Polizia stradale - e non solo - spesso costretta a non utilizzare le volanti a sua disposizione per mancanza di benzina oppure gli strumenti per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada, per fare solo alcuni esempi. Democratico, sulla quale si registrava in Commissione la convergenza di tutti gli schieramenti politici, e cioè quella di istituire un apposito fondo presso il Ministro dell'interno, con dotazione pari a 50 milioni di euro, da destinare all'acquisto e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di materiali, attrezzature e mezzi per lo svolgimento delle attività di controllo stradale, controllo stradale, nonché per le analisi cliniche e la ricerca e sperimentazione nel settore del contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, è stata respinta dal Governo con la motivazione della mancanza di risorse disponibili. Rimane del tutto incomprensibile come si voglia perseguire una maggiore sicurezza stradale senza prevedere un potenziamento, anche minimo, delle risorse a disposizione degli organi di polizia, drammaticamente ridotti nel corso degli ultimi anni e del tutto insufficienti alla missione loro assegnata. Altrettanto incomprensibili appaiono le posizioni assunte dal Governo in relazione alle varie proposte presentate dal Gruppo del Partito Democratico, mirate alla prevenzione e alla riduzione delle cause di maggiore incidentalità stradale. Fra queste si segnala la reiezione delle proposte innovative per una più efficace manutenzione ordinaria delle superfici stradali, per la realizzazione delle pavimentazioni delle superfici stradali e per l'installazione di nuove barriere di contenimento sulla rete stradale. Tali proposte nascono dalla lettura dei più recenti *report* statistici sull'incidentalità stradale diffusi dall'ISTAT e dalle forze dell'ordine, dai quali emerge in tutta evidenza che tra le principali cause di morte per gli utenti della strada, oltre alla distrazione, vi sono il cattivo stato di manutenzione e realizzazione della rete stradale

In terzo luogo, si lamenta il mancato accoglimento di alcune proposte mirate ad innalzare il livello di sicurezza e informazione degli utenti delle strade urbane ed extraurbane, con priorità per quelle a maggiore tasso di incidentalità. A tale proposito si segnala, solo per fare alcuni esempi, che il Governo ha posto il veto, sempre adducendo ragioni di bilancio, sulla proposta di potenziamento del servizio di infomobilità CCISS e Isoradio finalizzato ad aumentare la copertura oraria e territoriale del servizio offerto dai medesimi, al miglioramento della qualità di ricezione e per il rinnovo dei contratti e il potenziamento degli organici. Per non parlare, poi, della mancata approvazione della proposta per lo sviluppo dell'infomobilità finalizzata al sostegno di programmi di intervento predisposti da enti locali e dai proprietari e dagli enti concessionari delle predette strade, per garantire l'installazione e lo sviluppo di dispositivi di gestione informata della mobilità, di cartelli e dispositivi luminosi e di ogni altra strumentazione idonea all'informazione, in tempo reale, dell'utente delle strade. Sul tema dell'educazione alla guida è stato fatto lo stretto necessario e non si può non denunciare il mancato accoglimento delle proposte, il cui costo è estremamente ridotto, finalizzate alla predisposizione di apposite campagne di informazione per la conoscenza dei danni alla salute derivanti dal mancato rispetto delle regole di guida e per la realizzazione e diffusione di programmi finalizzati ad affrontare il problema della guida e degli incidenti stradali e a sostenere e coadiuvare i programmi di educazione alla guida. In conclusione, malgrado le criticità segnalate, il testo prodotto dalla Commissione e ora all'esame dell'Aula, nel merito e nel metodo, merita attenzione ed apprezzamento. Tra poco, in sede di dichiarazione di voto verrà definita la posizione del Partito Democratico, ma intanto vogliamo sottolineare che le norme che ci apprestiamo a votare ci fanno fare un passo in avanti. D'altra parte, questa è materia in continua evoluzione che ha la necessità di continue integrazioni alla luce del manifestarsi di comportamenti più o meno trasgressivi che producono insicurezza. Il Parlamento, troppo spesso, ha approvato provvedimenti tampone sulla scia di necessità immediate (si pensi solo come sul tema delle minicar in una settimana come sul tema delle minicar in una settimana si siano concentrate le attenzioni dei media e dell'opinione pubblica). Riteniamo, però, che provvedimenti "mordi e fuggi", se servono a dare risposte nell'immediato, rischiano di essere parziali e non pienamente efficaci. Per questo, auspichiamo che il tema della sicurezza stradale, da oggi in poi, sia oggetto di valutazione sistemica e che, dopo periodi più o meno brevi di sperimentazione di una normativa, si possa poi intervenire a ragion veduta sulla base di dati scientifici e di necessità reali e non perché piccoli gruppi di pressione sponsorizzano questo o quel provvedimento. Abbiamo sperimentato un metodo di lavoro che ci auguriamo anche per il futuro possa mettere al centro i problemi del Paese e dei cittadini prima che le identità partitiche, che pure vogliamo riconoscere come fondamentali per l'esercizio della democrazia.

il lavoro svolto in Commissione è stato importante, a dimostrazione della sensibilità su un argomento come questo, relativo alla sicurezza stradale. convinto che, alla fine, sia stato predisposto un buon testo, che sicuramente porterà maggiore sicurezza sulle strade, maggiori controlli e ci metterà in condizione di poter dire che siamo intervenuti per evitare ulteriori vittime della strada. Questo lo si è dovuto sicuramente al lavoro che

voi, qui in Senato, avete dimostrato che su provvedimenti di questo tipo è possibile aprire tavoli di mediazione. Spero che questo sia l'inizio di un rapporto diverso tra maggioranza e opposizione. La linea di demarcazione tra maggioranza e opposizione è giusto che ci sia, perché il consociativismo è

di un rapporto diverso su provvedimenti che non hanno colore politico ed interessano tutti cittadini. Anche per questo, ho voluto essere presente e ringraziarvi per il lavoro che tutti

di aver contribuito in pari grado a questo importante sforzo per raggiungere un obiettivo comune. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro,

In quella occasione il presidente Grillo ricordava i numerosi inviti e sollecitazioni ricevuti volti ad assicurare, badate bene, l'approvazione definitiva del disegno di legge in esame entro la pausa estiva: eravamo al 29 luglio, come dire che il passaggio al Senato poteva anche essere inutile. Su un quotidiano di ieri ci si chiedeva chi avesse vinto e chi avesse perso tra i portatori di istanze nel settore della sicurezza stradale. Questo è emblematico di come un tema fondamentale come quello al nostro esame rischi di essere banalizzato. La sicurezza stradale costituisce un problema assai complesso e multidimensionale caratterizzato da aspetti che vanno da quelli più propriamente demosociali (il numero di morti e di feriti e la gravità delle lesioni), a quelli di carattere culturale (la cultura della sicurezza stradale, l'informazione, la formazione, la comunicazione, la sensibilizzazione), per arrivare fino agli aspetti economici relativi alle risorse per garantire la stessa sicurezza. L'Italia, come gli altri Paesi dell'Unione europea, si era posta nel 2001 l'obiettivo di ridurre del 50 per cento il numero dei morti e dei feriti causati da incidenti stradali nel termine del 2010. Nel 2009 il nostro Paese ha centrato tale obiettivo. Purtroppo, però, dai primi dati raccolti dal Ministero dell'interno e dalla polizia stradale, nei primi tre mesi di quest'anno emerge una netta inversione di tendenza: la mortalità è tornata a salire, di ben il 17 per cento, e anche i feriti aumentano nuovamente rispetto allo scorso anno. Secondo i dati forniti, responsabili di questo inatteso salto all'indietro sarebbero le autostrade. Sorprendente e direi irresponsabile è parsa, all'Italia dei Valori, la proposta di innalzare il limite di velocità a 150 chilometri orari in autostrada. Ci siamo battuti affinché si eliminasse questa norma, che non avrebbe contribuito a formare un'etica della responsabilità specie tra i giovani. Vorrei sottolineare che senza dubbio vi sono delle parti del provvedimento sulle quali vi è stato un miglioramento rispetto al testo licenziato dalla Camera, che abbiamo contribuito a modificare e sulle quali certamente non vi poteva che essere una condivisione generale. Mi riferisco all'aumento delle sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista. che sia così che sia intensificato il giro di vite per chi modifica le ormai tristemente famose minicar, come è stato ricordato, attorno alle quali molti ancora sono i nodi da sciogliere e i problemi da affrontare. Ritengo inoltre importante anche il lavoro svolto dalla Commissione per prevedere l'impossibilità, per chi ha la patente sospesa, di guidare tali veicoli. Positivo è per noi il divieto di bere per i neopatentati, così come per coloro che sono in possesso di patenti professionali. Condividiamo l'inasprimento delle sanzioni per gli autotrasportatori che violino i turni di riposo, ma siamo contrari alle sanzioni da applicare a coloro che superino i turni di guida previsti, poiché troppo bassi, così come non concordiamo sull'innalzamento dell'età da 65 a 70 anni, dietro conseguimento di specifico attestato, della possibilità di guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati; siamo contro le deroghe. C'erano dei capisaldi in questo disegno di legge che avevano indotto qualcuno a dipingere la futura legge come quella della «tolleranza zero». Al di là dello *slogan* mediatico, è ovvio che, nonostante i tentativi fatti congiuntamente dall'opposizione, non è più possibile definirla in questo modo. È stato eliminato l'obbligo per i medici - introdotto alla Camera - di comunicare al Ministero dei trasporti alcune patologie dei loro assistiti.

È stata prevista la deroga di tre ore al giorno a chi si è visto sospendere la patente per guida in stato di ebbrezza, vanificando così di fatto il provvedimento. Le norme contro coloro che guidano in stato di ubriachezza, se non vogliono ridursi ad una presa in giro, devono essere dure e senza eccezioni. Non si tratta di essere illiberali, di introdurre soltanto divieti, si tratta piuttosto di anteporre il valore della vita, propria e degli altri, educando tutti ad un comportamento che aumenti la sicurezza complessiva. Non si può essere morbidi con chi guida ubriaco al volante. Basta tener presente, a questo proposito, il caso recentissimo dell'imprenditore di Melzo che, ubriaco, ha ucciso un'intera famiglia. Ebbene questa persona era un recidivo, si era già visto sospendere per due volte la patente. La sicurezza stradale non può essere certamente un fatto soltanto repressivo, punitivo, di inasprimento delle pene, ma deve consistere anche nella prevenzione, educazione, previsione e capacità di determinare alcuni fenomeni. Quando si parla di educazione alla legalità che a noi sta molto a cuore - si fa giustamente riferimento alle grandi questioni riguardanti l'usura, le varie forme di mafia, la produzione e lo spaccio di droga. Molto raramente si registra una percezione della pericolosità sociale dei comportamenti di guida che mettono a repentaglio non solo l'incolumità personale del conducente, ma anche di coloro che hanno la disavventura di trovarsi nella condizione di passeggeri o di terzi. Non riusciamo a spiegarci come si sia potuto procedere a sopprimere la previsione relativa all'educazione stradale nelle scuole, come si fa a non capire che il nodo centrale della sicurezza riguarda un fatto della massima importanza. Il rispetto della legge non può limitarsi all'area della repressione, ma deve essenzialmente riguardare la comunicazione delle motivazioni che sottostanno alla scelta normativa. La scelta del legislatore ha il compito precipuo di tutelare un bene, nel nostro caso il bene dell'incolumità e della vita in generale, ma tale scelta deve essere innanzitutto trasmessa. Sembra che la prevenzione sia un aspetto non importante della sicurezza. Cercare di evitare che le cose accadano è per noi invece fondamentale. Così si spiega, al di là delle sterili polemiche che l'hanno accompagnata, la nostra proposta emendativa sul divieto di fumo per chi è alla guida, trasformata in una "rondine" del giorno, Non si tratta, cari colleghi, di proibizionismo, ma solo di evitare che un calo del livello di attenzione mentre si guida possa provocare un incidente. Altri Paesi, senza dubbio più lungimiranti del nostro, come l'Inghilterra e la Svezia, lo prevedono già. Il nostro codice della strada dispone a sua volta che non possono essere usati apparecchi radiotelefonici mentre si è alla guida. Ci chiediamo prendere la sigaretta, accenderla e poi tenerla in mano mentre si guida, che differenza fa con il tenere tra le mani un cellulare e comporre un numero di telefono? Non è una banalità. Voglio aggiungere che la patente a punti ha portato una riduzione dell'incidentalità di circa il 20 per cento ma ha ormai esaurito l'effetto propulsivo: l'incidentalità ha ripreso infatti a crescere. Questo denota che tale modello va ripensato con un approccio diverso, ma certo non indebolito, come è avvenuto in questa

Non affrontare il problema della manutenzione delle strade equivale, se non stiamo attenti, a vanificare tutti gli sforzi di carattere legislativo sul tema. Le principali cause di incidentalità sono legate al comportamento umano, ma non esclusivamente a questo. Riteniamo positiva l'introduzione della destinazione, con precise percentuali e modalità, dei proventi degli autovelox tra Comuni ed enti proprietari delle strade. La sicurezza stradale può essere vista un po' come un sistema complesso, caratterizzato da diverse variabili. Si è affermato che la bicicletta è sia un mezzo di trasporto, sia un mezzo per il tempo libero. Non è un caso che, quando viene periodicamente diffusa la notizia relativa all'alto numero di morti tra ciclisti in Italia rispetto ad altri Paesi europei, l'unica indicazione che compare sulla stampa è l'invito ad utilizzare caschi e seggiolini omologati. Senza dubbio sono interventi utili, ma, dal punto di vista dell'efficacia, molti di tali interventi risponderebbero al problema della sicurezza solo se il ciclista non intersecasse mai il traffico Voglio concludere facendo soltanto un riferimento alla questione delle patenti dei conducenti delle famose auto blu. La nostra battaglia affinché venisse ritirato quell'emendamento non è stata vana. Ne abbiamo guadagnato tutti in termini di civiltà e di ricerca di un costume morale che ormai abbiamo perso. Per concludere, signor Presidente, mi rivolgo a tutti i colleghi e al Governo. Potevamo fare meglio invece abbiamo perso una buona occasione. Non si possono annunciare riforme e tagliare i finanziamenti. Senza soldi non si cantano messe, non si fa manutenzione stradale, non si fanno controlli sufficienti, non si fa prevenzione.

non può votare a favore del testo licenziato. Ci si augura che la Camera voglia porre rimedio ad alcune criticità che permangono e che abbiamo segnalato. Per tali motivi, il nostro Gruppo annuncia il voto di astensione. Presidente, onorevoli colleghi, ogni giorno in Italia si verificano in media 598 incidenti stradali. Nel 2008 4.731 individui hanno perso la vita 310.739 hanno subìto lesioni di diversa gravità. L'indice di mortalità mostra che gli incidenti più gravi avvengono nelle strade extraurbane e nei *weekend* e si mantiene superiore alla media nell'arco temporale che va dalle ore 21 alle 7 del mattino. I comportamenti errati di guida costituiscono le prime cause di incidente; tuttavia, lo stato psicofisico alterato del conducente va segnalato per la gravità degli eventi. La fascia più colpita dalle conseguenze degli incidenti stradali resta quella tra i 25 e i 29 anni. Ora, se è vero che in Italia tra il 2000 e il 2008 gli incidenti sono passati da 256.546 circa a 218.963, i i morti da 7.061 a 4.731, i feriti da 360.013 a 310.739, con una riduzione del tasso di mortalità dal 2,8 per cento del 2000 al 2,2 del 2008 e un indice di gravità dall'1,9 all'1,5 per cento di decessi per ogni 100 infortunati, il fenomeno si conferma in proporzioni comunque drammatiche. Nonostante il calo di incidenti, pari al meno 9,4 per cento siamo ancora lontani dall'obiettivo fissato dall'Unione europea nel Libro bianco del 2001, che prevedeva la riduzione della mortalità del 50 per cento Alla luce di questi dati, veramente tragici, dalla modifica delle disposizioni del codice della strada i cittadini si sarebbero aspettati risposte efficaci ai fini di tutelare la loro sicurezza sulle strade e la loro incolumità. Ma non vorrei che dovessero restare delusi da questo provvedimento, che si proponeva inizialmente un risultato ambizioso. Tuttavia, anche se alcune delle proposte avanzate appaiono condivisibili, il disegno di legge nelle sue articolazioni, così come è venuto fuori dalla Commissione in sede redigente, appare non all'altezza delle aspettative di quei cittadini e di quelle famiglie che reclamano tranquillità sulle strade per sé e per i propri figli. La sicurezza stradale non si realizza soltanto con la minaccia di una sanzione pesante finalizzata a far desistere i potenziali trasgressori dal porre in essere violazioni del codice della strada, ma anche con la predisposizione di un capillare sistema di controlli preventivi organizzati sull'intero territorio, la formazione degli utenti, soprattutto i più deboli, e una cultura diffusa della sicurezza. Se quindi alcune delle proposte contenute nel disegno di legge appaiono condivisibili, come dicevo, altre destano forti perplessità. Attraverso i nostri emendamenti, abbiamo sin da subito evidenziato quali dovessero essere le linee guida che avrebbero dovuto ispirare il provvedimento ovvero: miglioramento delle infrastrutture stradali e della segnaletica; sicurezza degli autoveicoli; controllo della condotta dei conducenti, con riferimento soprattutto ai neopatentati, alla popolazione anziana e, in particolare, ai casi di alterazione derivante dal ricorso ad alcol o droghe anche attraverso campagne di sensibilizzazione all'educazione comportamentale che incrementino la consapevolezza nella popolazione del rischio connesso all'uso di alcol e degli stupefacenti. L'abuso di alcol e sostanze, più in generale la cosiddetta cultura dello sballo, non solo del sabato sera, che coinvolge le fasce più giovani, con un rischio sempre maggiore di abbassamento dell'età, provoca infatti gli incidenti più eclatanti. Per questo vorremmo che si avesse il coraggio di fare di più; per questo ci siamo particolarmente battuti con un nostro emendamento al fine di vietare la somministrazione di alcolici e superalcolici nelle ore notturne nelle aree di sosta delle autostrade. La salvaguardia della vita dei più giovani, i più colpiti, e la difesa dell'integrità familiare rappresentano per noi un caposaldo da tutelare anche in questo contesto. Esprimiamo per questo un apprezzamento sull'introduzione dell'obbligo per chi chiede il primo rilascio della patente di guida nonché per chi chiede il rilascio del certificato di abilitazione professionale di produrre un certificato che attesti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti, nonché la previsione dell'obbligo dei sistemi di verifica del tasso alcolemico in tutti i locali ed esercizi pubblici abilitati alla vendita o alla somministrazione di bevande alcoliche. Non è accettabile che chi uccide guidando, in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di droghe, o semplicemente violando sfrontatamente le più elementari regole di sicurezza

che finisce per agevolare la condotta di colui che versa in questo stato piuttosto che aggravarne la responsabilità dolosa. Viene spontaneo chiedersi: è corretto considerare la criminalità "stradale" come sempre e necessariamente colposa? A questa domanda viene altrettanto spontaneo rispondere che noi siamo dalla parte della vita, sempre! In tal senso, abbiamo presentato un emendamento che si proponeva di ripristinare la facoltà di arresto in flagranza nei casi di omicidio colposo stradale, ma lo abbiamo trasformato in un ordine del giorno, considerando che non c'era la volontà di intervenire rispetto a norme contenute nel codice penale. Riteniamo altrettanto importante che di fronte a questo fenomeno, che purtroppo coinvolge soprattutto giovani e giovanissimi, si intervenga non solo in senso repressivo ma soprattutto preventivo e rieducativo. Per questa ragione, condividiamo la proposta che permette di accedere, in luogo della pena detentiva e pecuniaria, per una sola volta, per chi non ha provocato incidenti stradali, ma ha guidato sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti, al lavoro di pubblica utilità a favore della collettività da svolgere nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. La tutela dei più giovani e delle loro famiglie ci ha indotto a prestare particolare attenzione anche nei confronti dell'uso delle cosiddette minicar da parte dei giovanissimi. Troppo spesso un uso disinvolto e la mancanza di opportune regole di salvaguardia ha prodotto conseguenze drammatiche. Ed in virtù di un nostro emendamento è stato introdotto l'obbligo delle cinture di sicurezza. Sulla stessa scia si colloca l'inasprimento delle sanzioni per chi le utilizza con motori truccati e il divieto di salirvi a chi è stata ritirata la patente. Ci saremmo tuttavia aspettati maggiore attenzione per l'ammodernamento e la manutenzione della rete stradale, maggiori risorse per gli strumenti e il personale dedito ai controlli, maggior considerazione per la prevenzione a favore di una cultura della sicurezza stradale. La sicurezza, infatti, si realizza non solo aggiornando le norme del codice della strada, aumentando il presidio del territorio e l'adeguamento degli organici delle forze dell'ordine, al fine di individuare le responsabilità, punire gli autori con pene commisurate alla gravità dei reati ed assicurare alle vittime e ai loro familiari un risarcimento equo. La sicurezza si protegge inoltre con la formazione e la prevenzione. In tal senso ci saremmo aspettati - alcuni dei nostri emendamenti miravano proprio a questo - una maggiore attenzione riguardo alla concessione delle patenti di guida; la non conoscenza da parte dei candidati delle sanzioni cui andranno incontro violando le norme di legge per il comportamento alla guida, la loro ignoranza della gravità del problema e la mancanza di un serio accertamento tecnico in ordine alle caratteristiche psichiche dei candidati sono certamente tra le cause maggiori della incidentalità stradale. Così come maggiore attenzione si sarebbe dovuta riservare al rispetto dell'obbligo dell'educazione stradale. Comprendiamo l'esigenza della categoria degli autisti di rappresentanza; tuttavia non abbiamo assolutamente condiviso, in questa sede, l'emendamento a firma del senatore Gallo, che prevedeva la possibilità che gli stessi fossero esonerati dal rispetto delle regole di sicurezza, ritenendo piuttosto che fossero dotati di un'apposita patente professionale provvista di punteggio passibile di decurtazione. Condividiamo invece l'inasprimento delle sanzioni per gli autotrasportatori che violano le regole su tempi di guida e periodi minimi di riposo, ma non l'attenuazione dell'apparato sanzionatorio per le violazioni più lievi. Così come non abbiamo condiviso la possibilità, per i soggetti cui è stata sospesa la patente, di ottenere dal prefetto un permesso di guida speciale per determinate fasce orarie, né abbiamo condiviso l'innalzamento dell'età da 65 a 70 anni per i conduttori di scuolabus, TIR e per i cosiddetti padroncini. Questi ed altri dubbi ci hanno indotto a ritenere, fino alla fine, che ci fosse la necessità di una riflessione più approfondita che si dovesse svolgere in Assemblea. Il provvedimento, nella realtà, si è ridotto ad una visione abbastanza miope, che ricorre nella legislazione degli ultimi anni, consistente nella tendenza ad esaurire la capacità deterrente della norma nella sanzione (senza dubbio necessaria), trascurando la valenza preventiva ed educativa, che dovrebbe sempre accompagnare una produzione normativa lungimirante. Sebbene consideriamo questo provvedimento per certi aspetti positivo, crediamo che per altri aspetti si sarebbe potuto fare di più, procedendo in maniera differente, sia per l'*iter* legislativo che per ciò che riguarda le norme in esso introdotte. Avremmo voluto maggiori attenzioni e risposte alle richieste avanzate dall'Associazione nazionale delle vittime della strada. Abbiamo inoltre presentato un ordine del giorno sulla revisione delle norme di procedura penale. A nostro avviso, il rischio è di fare una riforma che non corrisponde alle aspettative e alle esigenze dei cittadini e che non aiuterà a colmare la percezione di divario fra il mondo reale e la politica.

Io credo che il lavoro svolto in questa Commissione sia stato certamente proficuo, interessante e collaborativo, da parte di tutti indistintamente. Il fatto che dal Ministero dell'economia sia giunto, soltanto all'ultimo momento, uno stop a quelli che potevano essere degli indirizzi molto più interessanti interessanti e più innovativi in un provvedimento del genere, soprattutto per ciò che riguarda l'aspetto della prevenzione e dell'educazione, ha reso veramente poco significativo nella sua *ratio* più generale il provvedimento, che pure era stato condotto a termine con tanta buona volontà e con la predisposizione, da parte di tutti, a conferire la sede redigente. che, se avessimo conosciuto le intenzioni del Governo per tempo, certamente non avremmo concesso la sede redigente ed avremmo dato all'Aula la possibilità possibilità di discutere maggiormente su contenuti di peso e fortemente innovativi. Il provvedimento, così com'è, non ci soddisfa assolutamente; il massimo dello sforzo di condivisione che possiamo fare è di dichiarare un voto di astensione.

come è stato ribadito dal relatore all'inizio, l'*iter* di questo provvedimento non è stato dei più agevoli. Si sono messi di mezzo le ferie, le fermate di lavori parlamentari, le elezioni, i pareri che certe volte non arrivavano, con il risultato che da parte dei colleghi dell'altra Camera, con il supporto di alcuni quotidiani, si è voluto quasi addebitare ai componenti della 8a Commissione del Senato una certa maggiore incidentalità sulle strade di conseguenza della non approvazione del provvedimento. Il problema della sicurezza stradale è stato sviscerato in tutte le sue sfaccettature con moltissime audizioni di tutte le componenti del settore e approfondendo ciascuno degli oltre 400 emendamenti presentati. Mi si permetta di ringraziare a tale proposito tutti i colleghi di Commissione che hanno saputo interpretare il lavoro comune senza assolutamente alcuna etichettatura di parte nonché il sottosegretario Giachino per la sua costante e competente presenza. L'ultima modifica del codice della strada è avvenuta nel 2007; dopo tre anni - giustamente - abbiamo rimesso mano, nella convinzione che quello della sicurezza stradale sia da considerarsi un problema aperto per il continuo divenire delle situazioni e perché certe norme hanno dei tempi di maturazione diversi. Sono dell'avviso che tra un paio di anni certi argomenti, che ancora oggi sono stati accantonati, verranno prepotentemente alla ribalta e si dovrà prenderli in considerazione anche perché penso che, almeno una volta, il legislatore dovrà anticipare la società, gettare le linee e non andare sempre a rimorchio. Qualche quotidiano, che mi sento di definire scandalistico, titolava a tutta pagina anche recentemente: divieto su divieto diventeremo schiavi. L'ultima follia: casco in bici per legge. Vorrei ricordare che tal Orietta B., di otto anni, morta battendo la testa per terra perché la gonna le si era avvolta tra i raggi della bicicletta, sarebbe ancora viva se avesse avuto la protezione del caschetto. Pertanto, ben venga il caschetto per i ragazzini fino a 14 anni. Una pubblicità che compariva sui giornali tedeschi quando ancora in Italia non era obbligatorio il casco per le moto diceva: se hai la testa, proteggila. Alla fine penso che sia una questione di maturazione sociale che spetta al legislatore coltivare, anche perché un infortunio,

per coloro che si sono visti ritirare la patente per varie motivazioni. Si tratta di ore di permesso di guida che verranno recuperate raddoppiandole con un allungamento della sanzione, come suggerito magistralmente dal nostro collega di partito, senatore Vallardi. La lega Nord, con alto senso di responsabilità, al fine di non frapporre ostacoli all'assegnazione in sede redigente del provvedimento, non ha insistito sull'elevazione da subito a 150 chilometri all'ora del limite di velocità su quei pochi tratti autostradali a tre corsie, più quella di emergenza, e muniti di *tutor*, che pur aveva avuto il parere favorevole da parte del Governo, che annualmente, in sede di verifica da parte del proprietario e concessionario dell'autostrada, sia esaminata la fattibilità di un innalzamento del limite ricorrendo tutte le situazioni di sicurezza prevista, attuando, in buona sostanza, quanto già previsto nel testo di legge. Questi sono soltanto alcuni esempi di quanto è stato inserito in questo disegno di legge e che la Lega Nord ha convintamente sostenuto.

pareggiando in questo modo il rispetto che noi abbiamo avuto per il testo arrivatoci dalla Camera dei deputati; ciò al fine di non arrivare ad un infinito «palleggiamento» tra Camera e Senato. Pertanto, annuncio a nome del Gruppo della Lega Nord Padania il voto favorevole a questo provvedimento.

per un atto - voglio dirlo subito, a scanso di equivoci - risultato alla fine distante non solo dai nostri desideri, ma anche dalle attese suscitate nel corso dei lavori e dalle reali possibilità che sarebbe stato ragionevole cogliere con il lavoro prodotto in questi mesi. Ci siamo adoperati in maniera intensa, con spirito costruttivo e con sincera generosità, perché sappiamo che dalla mancanza di sicurezza sulla strada deriva per il nostro Paese un tributo insopportabile in termini di vite umane, di fronte alle quali non c'è per quanto nobile - alcuno spirito di parte che tenga. Per questo non abbiamo tollerato banalizzazioni, strumentalizzazioni e speculazioni al limite della volgarità, veri e propri atti di sciacallaggio su sciagure che hanno segnato e che purtroppo ogni giorno segnano irrimediabilmente vite e relazioni umane, e che da parte di autorevoli esponenti delle istituzioni - lasciatemelo dire avrebbero richiesto maggiore compostezza e, di certo, maggiore senso di rispetto per il dolore umano. Vede signor Ministro, non siamo usi a raccontarci barzellette su temi di così grande delicatezza. verificata invece, come il sottosegretario Giachino sa bene per aver seguito in maniera encomiabile tutti i lavori della nostra Commissione, la disdicevole situazione per cui, mentre si interveniva per modificare il provvedimento con significativi emendamenti proprio sul tema delle minicar, abbiamo vissuto la sgradevole sensazione che si volesse gettare discredito un lavoro che era teso non a stravolgere il provvedimento licenziato dalla Camera, ma semplicemente ad apportare i miglioramenti necessari. Questo, soltanto questo, è stato il nostro obiettivo nei defaticanti lavori della Commissione, i cui numeri, che sono stati già rappresentati molto bene dai relatori, probabilmente non danno la cifra esatta dell'impegno e del clima che si è realizzato intorno a questo provvedimento, di cui do volentieri atto al Presidente della Commissione, senatore Grillo, e al relatore, Ho voluto fare questa premessa perché per noi, voglio essere chiaro signor Ministro, sarebbe stata più opportuna - pensi un po' - anziché una legge di iniziativa parlamentare, una legge delega al Governo per la riscrittura del codice della strada e ciò per alcuni essenziali motivi che voglio esporre. In primo luogo perché nel tempo il codice della strada ha subito tanti e tali rimaneggiamenti da essere di fatto divenuto incomprensibile perfino agli stessi cultori della materia; e ciò è tanto più paradossale proprio in ragione del suo indiscusso valore di uso quotidiano per milioni di cittadini. La riscrittura del codice della strada, in secondo luogo, si sarebbe resa necessaria, a nostro avviso, anche per dare al codice una struttura più flessibile,

era necessario un lavoro, da parte del Parlamento, più cogente sul piano degli indirizzi, in specie di quelli inerenti alla sicurezza stradale, in termini di obiettivi e di strategie sottese. Un lavoro tanto più opportuno proprio perché ci troviamo alla vigilia di una fase in cui saremo chiamati a fare un bilancio di una stagione in cui, per tutti i Paesi membri, gli obiettivi fissati dall'Unione europea per il 2010 prevedevano - come sappiamo e come è stato ricordato - il dimezzamento nel decennio delle vittime per incidenti stradali. Tale obiettivo non è stato conseguito e ciò nonostante negli anni siano state fatte cose apprezzabili, tanto dai Governi di centrodestra quanto da quelli di centrosinistra, che negli ultimi anni ci hanno visto concorrere nei provvedimenti sulla sicurezza stradale sostanzialmente in maniera condivisa pur partendo da ispirazioni culturali profondamente diverse. Il nostro Paese si ferma, per il 2009, al 33 per cento di riduzione delle vittime della strada, lontano da Paesi virtuosi come Portogallo e Lussemburgo, che hanno raggiunto l'obiettivo di riduzione del 50 per cento con un anno di anticipo, ma anche da Paesi con i quali il raffronto,

Le ragioni di questo ritardo, per chi vuole uscire da un approccio emotivo e - mi sia consentito - talvolta "spannometrico", sono purtroppo impietose, tanto sul piano dei controlli stradali effettuati, quanto su quello delle risorse impiegate per migliorare l'infrastruttura stradale, aspetti che avrebbero dovuto invece qualificare il provvedimento in esame. Da questo punto di vista, i dati dimostrano che il nostro Paese, mediamente, fa circa un decimo di ciò che i Paesi più virtuosi realizzano, e comunque in misura sensibilmente inferiore alla media europea.

chiari anche il contesto in cui questi incidenti prevalentemente si consumano e le principali cause. Il contesto è quello urbano, soprattutto nelle nostre città di medie e grandi dimensioni; ciò a causa della più alta intensità di traffico, ma anche per il peggiore stato delle manutenzioni delle infrastrutture stradali: assenza di manti drenanti e segnaletica inadeguata. Di evidenza solare, purtroppo, è anche che la prima causa di morte negli incidenti stradali è costituita dalla velocità, che riduce i tempi di reazione, allunga talvolta inesorabilmente i tempi di frenata e presuppone sempre un controllo più vigile della guida,

Recentemente, un mio caro amico, padre di una giovane quattordicenne, mi ha confessato disarmato di vivere nell'angoscia di un genitore che è consapevole di avere la propria figlia in guerra. Il bollettino quotidiano dei caduti e dei feriti che ogni giorno si consuma, del resto, è eloquente. Ed allora la sicurezza non la si può ottenere soltanto inasprendo le sanzioni, che di per sé non sono in grado di costituire il sufficiente deterrente ai comportamenti di guida pericolosa. Molti dei messaggi che sono stati veicolati come un mantra dai media in questi mesi hanno affermato la necessità di adottare provvedimenti a tolleranza zero. Signor Ministro, mi permetto di ricordare innanzitutto a me stesso che Rudolph Giuliani,

nella difficoltà di passare da una cultura degli atti ad una cultura dei fatti, in grado di produrre cambiamento vero, nelle cose ma anche nella cultura di un Paese. in questo provvedimento, alla fine, siano mancati proprio gli obiettivi che potevano essere più qualificanti, in termini di maggiori controlli stradali, ma anche di finalizzazioni certe dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in investimenti nelle infrastrutture, come prevedeva il provvedimento approvato alla Camera. Adesso il rischio più grosso è quello di avere prodotto norme manifesto, buone certo per "editti di carta", meno per conseguire quegli obiettivi ambiziosi e giusti che in sede comunitaria ci adoperiamo e concorriamo a definire. Piuttosto abbiamo avvertito, anche in questo provvedimento, l'invalsa convinzione da parte del Governo che sia possibile fare riforme vere senza risorse. Voglio dirlo nella maniera più semplice: non è possibile! Badate che non siamo così sciocchi o incoscienti da non capire la situazione che stiamo attraversando. Il punto, però, è un altro: non si può pretendere di innovare, di voler introdurre processi di cambiamento ritenuti necessari essendo al contempo conservatori dell'esistente. Se non vi sono risorse aggiuntive (come è evidente), il cambiamento si produce ottimizzando quelle esistenti; per farlo, però, occorre scegliere e sfidare il consenso, cosa che - nonostante i vostri proclami - non siete più in grado di fare. Soprattutto la cosa più odiosa è che anche per la sicurezza stradale non si può ricorrere, con tanta disinvoltura, soltanto al portafoglio dei contribuenti. Così facendo, si produce solo distanza e disaffezione. Ecco, noi abbiamo voluto dimostrare e dimostrarvi che anche in momenti difficili per il Paese si possono assumere scelte di responsabilità nell'interesse della collettività, dopo aver contribuito a migliorarle, ovviamente dal nostro punto di vista. Rivendichiamo per intero la nostra autonomia di giudizio che, su questo provvedimento, non può essere in sintonia con la vostra, come avremmo invece voluto che fosse e come abbiamo fino da ultimo cercato di perseguire. Per questo motivo, il nostro sarà un voto di astensione sul provvedimento. In ultimo, signor Ministro (mi sia concesso ancora un minuto di tempo), mi rivolgo direttamente a lei. Si è parlato nelle ultime ore di un possibile decreto ministeriale se non fosse stata accolta la sede redigente. Non so e non mi interessa sapere se questa voce sia corrispondente al vero. che, se ciò fosse stato fatto, avrebbe avuto il significato politico di mettere in scacco il Senato e forse anche l'intero Parlamento nella sua presunta incapacità di decidere, nelle fasi complesse, in tempi ragionevoli per l'interesse del Paese e dei cittadini. Voglio affermare tranquillamente che non abbiamo avvertito questa eventualità come una minaccia o un ricatto. Adesso, però, sta anche a lei scortare questo provvedimento,

Prima di motivare in modo sintetico le ragioni di questo voto, desidero ringraziare in primo luogo il signor ministro, senatore Altero Matteoli, per l'impegno profuso seguendoci quotidianamente e per la disponibilità offerta suoi Uffici a collaborare in maniera continuativa con la Commissione; ringrazio altresì il sottosegretario Giachino per la sua quotidiana presenza, che ha sottolineato una continuità da parte del Governo nei lavori della Commissione.

di una revisione organica e puntuale del codice della strada, che si muovesse lungo una linea di coerenza verso l'introduzione di norme ancora più severe rispetto a quelle esistenti.

hanno tentato di addossarci responsabilità che riteniamo di non avere. A coloro che hanno lamentato i tempi troppo lunghi nel predisporre questo provvedimento, abbiamo spiegato che si è trattato di un lavoro complesso, com'è stato ricordato anche dal relatore, che ha richiesto quotidiane verifiche tecniche su materie regolamentate da direttive europee, da norme nazionali, da regolamenti di esecuzione e da circolari interpretative. Qualcuno, signor Presidente, con un'evidente caduta di stile che si commenta da sé, nel criticare questa lunghezza dei tempi, che certamente c'è stata, ha perso il senso della misura, arrivando a criticare addirittura il bicameralismo in quanto tale. In questo modo si sono date in pasto all'opinione pubblica del nostro Paese affermazioni del tutto gratuite, del tipo: «Mentre i senatori discutono se è possibile fumare in auto, aumentano i morti sulla strada!». Ha ragione il senatore Filippi: abbiamo assistito ad episodi di sciacallaggio davvero inauditi. A queste provocazioni comunque, come maggioranza e minoranza, abbiamo risposto e rispondiamo esibendo la positività di un risultato politico che oggi in Aula fa registrare con grande soddisfazione una posizione in qualche modo condivisa, perché l'opinione dominante è quella di avere un testo che migliora quello esistente e che perfeziona il lavoro fatto dai colleghi della Camera. Un lavoro politico, dunque, che dimostra semmai

Consegniamo quindi ai colleghi della Camera un testo migliorato in ben 60 articoli, che abbiamo riformato muovendoci fondamentalmente lungo tre linee di lavoro.

che apparivano a tutti fin troppo evidenti nella valutazione svolta dall'altro ramo del Parlamento. Per un altro verso, abbiamo dovuto coordinare il nuovo testo con le leggi nel frattempo approvate dal Parlamento e con la legge n. 94 del 2009 sulla pubblica sicurezza. Per un altro verso ancora, l'intelligenza di tutti noi ci ha spinto a produrre nuove norme, frutto di suggerimenti avanzati da enti ed associazioni che abbiamo

Ritengo di non dover rispondere a tutte le questioni che ci ha già ricordato il senatore Cicolani. Mi limiterò soltanto a sottolineare due Il primo è che la trama del lavoro politico che oggi si conclude ha una sua coerenza: lo abbiamo voluto con forza. Le modifiche, cioè, rispondono e questo è inconfutabile, nonostante ciò che scrivono taluni distratti giornalisti, commentatori di questi temi - ad una linea che la Commissione ha fatto propria: introdurre istituti nuovi e norme più severe per garantire concretamente più sicurezza sulle strade italiane. Potevamo fare di più? Probabilmente. Ciò che non siamo riusciti a normare lo abbiamo lasciato all'attenzione del Governo in sede di proposte e di ordini del giorno. Ma la questione

e dalla senatrice Poli Bortone che, nell'ultima parte del suo intervento, ha ricordato il ruolo della Ragioneria generale dello Stato) è la cosiddetta questione delle risorse.

di un ruolo preponderante da parte del Ministero dell'economia, quindi degli apparati che supportano la linea politica del Ministero, che decide che decide e condiziona sempre di più la produzione legislativa di questo Parlamento. Ritengo che questo sia giustificato dall'emergenza nella quale ancor oggi si trova il nostro Paese: un'emergenza che - dobbiamo il Governo ha affrontato con una politica di rigore economico che finora ha consentito al Paese di reggere e di non entrare nella zona buia dei Paesi in qualche modo fragili

burocraticamente eccellenti, senz'altro assai qualificati - potessero mettere in discussione la libertà del Parlamento di produrre nuove norme e di attestare le risorse a sostegno delle stesse in modo diverso da come, a legislazione vigente, ci è dato di apprendere. Ma questo è.

ma pensi anche che nella concorrenza globale: nella società globalizzata, la competitività è la regola con cui un Paese sta o non sta sul mercato, sta o non sta o non sta nelle condizioni di reggere la concorrenza che arriva da tutti gli altri Paesi. E allora, in questo senso, anch'io auguro che arrivi presto questa seconda fase, che si riaprano i cordoni della borsa e si metta in conto di fare una politica mirata più alla crescita che all'obbedienza cieca di parametri che, anche a mio modo di vedere, sono superati ancorché oggi siano utili a mantenere la barca in equilibrio.

al voto. Non potrei naturalmente votare contro, perché il provvedimento contiene molte norme importanti per la sicurezza stradale, e sono grato dell'encomiabile lavoro dei colleghi, in particolare del mio Gruppo. Del resto, l'ampio consenso che il provvedimento ha conseguito mi consente di segnalare in modo solitario una questione. È l'impianto generale del provvedimento che non mi convince: nuovi oneri, nuovi divieti, nuovi obblighi. Lo Stato non è in grado di far rispettare quelli esistenti e noi ne aggiungiamo di nuovi, pensando di adempiere ad un nostro dovere: ma questi resteranno inadempiuti come gli altri, e non ne valutiamo sufficientemente l'effettiva necessità e realizzabilità. Faccio solo un esempio: si obbligheranno tutti i pubblici esercizi a dotarsi di un etilometro, obbligo già previsto nei grandi esercizi come le discoteche, in cui si va a bere, si va a bere molto e purtroppo anche a consumare altre sostanze. Sono serviti a poco o nulla. Adesso, con queste norme, anche l'ultimo bar dell'ultimo paesino d'Italia, dove si trovano i tre pensionati a giocare a carte e a bere, come si dice dalle nostre parti, un'«ombra», un bicchiere di vino, dovrà avere l'etilometro e un adeguato spazio di riposo. Nessuno utilizzerà questo etilometro, però i produttori di etilometri avranno un bel vantaggio! Nessuno lo utilizzerà, perché questo succede nelle discoteche. Ma perché esercizi, microimprese, oberate da una congerie di norme fiscali, sanitarie e autorizzative devono farsi carico anche di questo? Chi è attento, cari colleghi, o non beve o si è comprato l'etilometro e lo tiene in macchina. Perché dobbiamo prevedere in tutta Italia etilometri che resteranno in un angolo di questi esercizi, inutilizzati? Dobbiamo avere, cari colleghi, più fiducia nei cittadini e nella promozione attiva di comportamenti responsabili: non moltiplicazione di obblighi o divieti, ma collaborazione. Con un piano concordato con i pubblici esercizi, invece di norme superflue, si otterrebbe molto di più. O con un piano organizzato con le associazioni rappresentative dei ciclisti: invece del casco obbligatorio per legge, che per fortuna è stato corretto, era l'occasione per approvare i disegni di legge dei colleghi della maggioranza e dell'opposizione che prevedono più piste ciclabili, più itinerari ciclabili in campagna, più aiuti per le campagne delle associazioni ciclistiche e per l'adozione di comportamenti virtuosi. In In questo modo si ottengono risultati concreti e duraturi, che camminano sulle gambe di una convinzione collettiva piuttosto che su quelle un po' pretenziose, cari colleghi, di uno Stato regolatore di ogni comportamento umano.

deputati è intervenuta sugli articoli 17, in misura di mero coordinamento tecnico, 20, 30, 31, 32 e 50. Già in Commissione lavoro si è ritenuto opportuno, con un voto conforme, di mantenere nell'esame da parte del Senato la medesima perimetrazione realizzata alla Camera. *(Brusio).* PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Castro. Colleghi, Colleghi, per cortesia, è una discussione rapida e limitata; ciononostante se si potesse

*relatore*. Dicevo dunque come la Camera abbia limitato il proprio esame ed il proprio intervento agli articoli 20, 30, 31, 32 e 50, intervenendo con una norma di mero coordinamento sull'articolo 17. Conformemente a quanto deliberato dalle Commissioni riunite del Senato nei giorni scorsi, chiedo che l'Aula confermi la medesima perimetrazione dunque chiedo che l'esame del disegno di legge sia limitato: all'articolo 20, che dispone l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge n. 51 del 1955; all'articolo 30 in materia di clausole generali e di certificazione del contratto di lavoro; all'articolo 31, che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro; all'articolo 32, che concerne decadenza e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e all'articolo 50, che contiene invece disposizioni in materia

Signora Presidente, colleghi, è ovvio che nella discussione odierna non si può non partire dal messaggio del Presidente della Repubblica. Sulla base di esso la Camera dei deputati ha ritenuto di dover intervenire solo su cinque articoli del cosiddetto collegato lavoro. Credo che questa scelta, pur certamente legittima, sia errata e non possa essere condivisa da questo ramo del Parlamento, perché nasce da un'interpretazione eccessivamente restrittiva proprio del messaggio presidenziale. Il giudizio negativo del Capo dello Stato, se si appunta in particolare sugli articoli 20, 30, 31, 32 e 50 del provvedimento, non si limita però a essi ma investe l'intero provvedimento e questo sia nel merito che nel metodo. Da un lato, viene infatti stigmatizzata l'estrema eterogeneità di tutto il provvedimento, dall'altro viene sottolineata la criticabile tendenza a legiferare con provvedimenti *omnibus*. Come sottolineato dal Presidente, l'eterogeneità, la lunghezza e la complessità del testo hanno effetti negativi sulla comprensibilità delle disposizioni, sull'organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto. Originariamente il provvedimento, nato dallo stralcio di un provvedimento collegato alla finanziaria del 2009, avrebbe dovuto essere una delega al Governo per la riorganizzazione della normativa in tema di lavoro pubblico e privato, lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi aspettative e permessi, lavoro sommerso, controversie di lavoro, ammortizzatori sociali. Nel corso delle varie letture parlamentari sono state via via eliminate tutte le principali e più controverse disposizioni in tema di lavoro e in particolare quelle sulla mancata regolarizzazione dei precari nella pubblica amministrazione, che il ministro Brunetta ha preferito inserire in un provvedimento *ad hoc*. Ricordo che inizialmente il provvedimento si componeva di soli nove articoli, ma nel corso del suo lunghissimo e travagliato *iter*, iniziato il 5 agosto del 2008, è stato gonfiato ad opera del Governo e della maggioranza fino a contare ben 50 articoli sulle materie più disparate, dalle disposizioni sul *doping* a quelle in tema di sanità, dalle elezioni universitarie ai trasferimenti dei ricercatori, dalle norme sulla *privacy* in materia di di notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chi è addetto ad una funzione pubblica a quelle sulle vaccinazioni obbligatorie. Il risultato è, come sottolineato dal Presidente della Repubblica e già denunciato da noi dell'opposizione in precedenti passaggi parlamentari, un provvedimento in cui, accanto a norme avulse dall'oggetto del provvedimento e dal contesto in cui sono inserite, la normativa e le deleghe al Governo in tema di lavoro costituiscono solo una minima parte dell'insieme. Per quanto peraltro concerne nello specifico questa materia, non si può assolutamente condividerne il merito.

deleghe che significano l'espropriazione del Parlamento e della sua funzione legislativa su materie di importanza capitale nell'attuale momento di crisi economica e sociale. l'attenuazione delle sanzioni contro il lavoro sommerso, le modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro, la disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, normativa in materia di aspettativa dei dipendenti pubblici, la modifica alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap. E poi le norme sul contratto di apprendistato, che hanno costituito (lo ricordiamo benissimo tutti), insieme all'arbitrato, l'oggetto di più aspro dibattito nel corso dell'ultimo passaggio parlamentare del «collegato lavoro». Una pessima norma con cui si abbassa il limite scolastico obbligatorio, attualmente di sedici anni, consentendo, a chi lo volesse, di iniziare a lavorare come apprendista già a quindici Una disposizione controcorrente rispetto all'orientamento dell'Unione europea e che rischia di innalzare ulteriormente i livelli di abbandono scolastico in Italia. E ancora, l'uso strumentale delle norme sulla certificazione del contratto di lavoro. Ed infine, il famigerato articolo 31, l'introduzione dell'arbitrato obbligatorio in materia di controversie individuali di lavoro, su cui non a caso in particolare il presidente Napolitano punta il dito. A tale proposito sono certamente da valutare in maniera positiva le modifiche apportate alla Camera dei deputati, tuttavia ci sarebbe ancora molto da fare per migliorare l'articolo. Purtroppo, l'orientamento del Governo, a leggere le dichiarazioni di vari suoi esponenti, sembra essere esattamente l'opposto: la volontà di deregolamentare la materia del lavoro e dei contratti, nella logica di un incontro cosiddetto libero delle forze del lavoro nell'ambito del mercato. Ma il rafforzamento e la valorizzazione dell'autonomia delle parti non fa i conti con la diversità delle parti stesse; non si garantisce, infatti, la parte più debole, ovvero il lavoro e colui che fornisce il lavoro, ma è favorita ancora una volta l'azienda, proprio perché ha di fronte degli interlocutori deboli. La drammatica attuale situazione del lavoro in Italia, caratterizzata dalla presenza dì un vero e proprio esercito di lavoratori precari, richiedeva e richiede ben altro approccio e ben altre soluzioni. Riesaminando l'intero testo potremmo, per esempio, rivedere i tempi della riforma degli ammortizzatori sociali, per i quali invece è stata prevista una ennesima proroga. Questo l'invito che a nome del Gruppo Italia dei Valori rivolgo a tutta l'Assemblea: se vogliamo davvero rendere un servizio al Paese e rispondere realmente ai rilievi del presidente Napolitano, allora che il voto di questa Assemblea sia a favore della ridiscussione nella sua interezza del collegato lavoro. Signora Presidente, colleghi, il Gruppo del Partito Democratico si è espresso negativamente in Commissione e intende ribadire ora la propria contrarietà alla proposta del relatore di limitare l'esame del provvedimento ai soli articoli già esaminati e modificati alla Camera. Le ragioni di questa contrarietà sono molte e, innanzitutto, sono rinvenibili, come è stato detto dalla collega, nel messaggio motivato con cui il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere per una nuova deliberazione il provvedimento. Vale la pena ricordare che questo evento accade per la prima volta dall'inizio di questa legislatura: è la prima volta che il Presidente utilizza questo potere straordinario conferitogli dalla Costituzione. Nel proprio messaggio il Presidente richiama puntualmente l'*iter* parlamentare della legge, mettendo in evidenza il "travaglio" che l'ha caratterizzata e che ha portato, dopo oltre diciotto mesi di discussione, all'approvazione di una legge di straordinaria ampiezza e complessità. Vale ricordare che, nel corso dell'*iter*, sono stati espunti dal testo, anche grazie alla discussione parlamentare, numerosissimi altri articoli inerenti le materie più disparate, ma che sono ancora presenti numerosi articoli (ne abbiamo individuati tredici!) il cui contenuto non è coerente con la rubrica del provvedimento, con le materie del lavoro e con le competenze delle Commissioni chiamate a svolgere in sede referente l'esame del provvedimento. Un esempio per tutti: ben cinque articoli, dall'8 al 12, intervengono regolando questioni attinenti il personale universitario e sulla riforma dell'università è in corso, proprio presso la Commissione Senato, la discussione di un testo di riforma. Non capiamo quale sia la logica in ragione della quale si separa e si disperde la discussione e la deliberazione sulla medesima materia, con risultati certamente disorganici e di cattiva legislazione. È proprio sul tema della cattiva qualità della legislazione che mi vorrei soffermare. Il presidente Napolitano rimarca come la «marcata eterogeneità» del provvedimento delimiti un modo di legiferare, più volte censurato anche dal nostro Gruppo qui al Senato, con interventi e documenti e con una mozione; una modalità che «mina la certezza del diritto», rendendo le leggi non conoscibili e non comprensibili in piena violazione del principio democratico. Non si tratta di un rilievo marginale: non assumerlo come guida del riesame del provvedimento, limitando l'esame ai soli cinque articoli esplicitamente oggetto di osservazione significa andare verso un indebolimento della presunzione di conoscenza delle leggi e del, conseguente, dovere di rispettarle. Si può, inoltre, facilmente prevedere il fiorire di esercizi interpretativi e lo sviluppo esponenziale di quel contenzioso, la cui deflazione appare tra gli obiettivi espliciti del provvedimento, con conseguenti costi suppletivi per lo Stato, per i cittadini e per le imprese. Ci sembra strano non riscontrare questa sensibilità in un Governo e in una maggioranza che hanno fatto della semplificazione e della sburocratizzazione una bandiera, propagandata ogni giorno e con ogni mezzo. Una legislazione oscura, non esplicita, non accessibile è la rappresentazione più chiara della lontananza delle istituzioni dai cittadini e del venir meno della loro legittimità democratica. Questo è tanto più vero quando, come ricorda il Presidente, i «provvedimenti legislativi» siano «relativi a materie di particolare rilievo e complessità» e «disciplinino temi di indubbia delicatezza sul piano sociale, attinenti alla tutela della salute e di altri diritti dei lavoratori». II presidente Napolitano ci consegna l'occasione - preziosa e non ricusabile - di svolgere al meglio il nostro lavoro, riconsiderando il provvedimento nella sua totalità, migliorandone la qualità sia redazionale che di contenuto. Se non lo faremo avremo sprecato un'occasione preziosa e l'auspicio del Presidente sarà caduto nel vuoto. Non farlo significa non cogliere l'opportunità di riconsiderare temi di grande rilevanza, soprattutto in riferimento alla grave crisi economica ed occupazionale che l'Italia sta attraversando. In questa fase il disegno di legge "lavoro" avrebbe dovuto essere, dovrebbe essere una grande legge di riforma del mercato del lavoro, degli strumenti per proteggerlo, promuoverlo, qualificarlo, accompagnarlo attraverso la crisi e verso il suo superamento. Si muove invece su tutt'altri binari: quelli della destrutturazione

Non tutte le criticità segnalate dal Capo dello Stato sono state risolte: auspichiamo che nella lettura al Senato si possa procedere al miglioramento del testo affermando soluzioni più semplici e nette, di piena coerenza del testo con i princìpi costituzionali e con le disposizioni di legge che tutelano i diritti costituzionali e fondamentali dei lavoratori, distinguendole dalle materie regolate dalla contrattazione collettiva, sulla cui regolazione anche in presenza di contenzioso le parti sociali devono essere sovrane. Ma vi sono nel testo numerose altre previsioni che destano grave preoccupazione e che meritano di essere ridiscusse. Le cito rapidamente (le ha ricordate anche la collega che mi ha preceduto). Si tratta dell'ulteriore dilazione dei termini di esercizio della delega sui lavori usuranti; dell'ulteriore differimento dell'esercizio della delega sulla riforma degli ammortizzatori sociali e sulle riforme per favorire l'occupazione femminile; del ridimensionamento delle procedure e delle sanzioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso; della revisione delle norme in materia di orario di lavoro, che - fra l'altro - hanno aperto la strada alla possibilità di ammettere ai negoziati e agli accordi derogatori dei contratti collettivi sigle sindacali con esclusiva rappresentatività territoriale; territoriale; di molte norme che penalizzano particolarmente le lavoratrici, fra cui quella sulla revisione dei contratti *part-time* nella pubblica amministrazione; da ultimo, ma non ultimo per importanza, si tratta di un intervento di inusitata gravità, quello dell'articolo 48, comma 8, in base al quale si prevede che l'ultimo anno dell'obbligo di istruzione possa essere assolto «anche nei percorsi di apprendistato», abbassando di fatto a quindici anni l'età di accesso al lavoro. Per tutte queste ragioni, ribadiamo la nostra totale contrarietà a limitare l'esame ai soli articoli proposti dal relatore e invitiamo la maggioranza a rivedere la propria decisione, ormai non più sostenuta nemmeno dall'obiettivo di giungere rapidamente all'approvazione definitiva del testo: infatti sono già state annunciate modifiche al testo dei cinque articoli oggetto dell'esame presso la Camera, che imporranno naturalmente un'ulteriore lettura, dopo la lettura del Senato, da parte della Camera stessa. Non c'è quindi un fattore tempo a sollecitarci. Auspichiamo che si tratti di interventi rispettosi dei miglioramenti prodotti dalla discussione parlamentare e delle sollecitazioni pervenute dal Capo dello Stato e non di mere riproposizioni della visione unilaterale del Governo. E d'altro canto, e da ultimo, il disegno di legge sarà nuovamente votato - articolo per articolo e poi nel suo complesso, come prevede l'articolo il comma 2 dell'articolo 136 del nostro Regolamento - giungendo ad una nuova deliberazione complessiva. Non si vede quindi nemmeno da questo punto di vista per cui, se il testo deve essere integralmente rivotato, l'esame e la discussione debbano essere limitati ai soli cinque articoli indicati dal senatore Castro. È più che mai importante che il Parlamento si dimostri all'altezza del compito e intervenga legiferando nell'interesse dei lavoratori tutti e dei cittadini, con la trasparenza e la ponderazione necessarie. Gli strumenti e il tempo ci sono; occorrerebbe la volontà di farlo.

il presente disegno di legge - com'è stato ricordato - ha avuto una vita travagliata. Nato con pochi articoli, man mano ha ricevuto una sorta di implementazione che l'ha portato alle dimensioni che tutti quanti conosciamo. Siamo ormai in sesta lettura e le vicende sono note. In data 31 marzo 2010 il Presidente della Repubblica, con un messaggio diretto alle Camere, ha rilevato una serie di osservazioni, in modo particolare dubitando della costituzionalità (anche se non in maniera abbastanza chiara e specifica) specifica) di alcune questioni. Egli ha fatto anche un discorso di carattere generale in ordine alla tecnica di legiferazione, che non è un problema recente, ma è un problema ormai noto, sul quale più volte le due Camere si sono soffermate, e riguarda la chiarezza e l'omogeneità delle materie trattate e la uniformità di tutto il provvedimento. Si sa bene che il dibattito parlamentare spesso spazia, si amplia e necessariamente porta a far diventare più vasto il bacino di discussione della legge stessa, così come è accaduto in questo caso. Il disegno di legge è già stato esaminato dalla Camera, dove sono state apportate determinate modifiche; indubbiamente i rilievi e le osservazioni mossi dal Presidente sono stati tutti presi in considerazione. I punti focali sui quali maggiormente si è accentrata l'attenzione del Presidente della Repubblica riguardavano in modo particolare l'arbitrato. Si è detto che lo strumento certamente non consentiva la difesa del lavoratore, soprattutto nel momento delicato della costituzione del rapporto di lavoro, e che poteva riguardare anche un altro momento delicato: quello della risoluzione del rapporto di lavoro.

successivo all'espletamento del periodo di prova e quindi garantiscono il lavoratore nel momento in cui il rapporto si consolida e diventa definitivo; esse non offrono quindi spazio a quelle titubanze e a quelle debolezze che forse giustamente sono state richiamate. È stato indicato anche un principio che ci sembra molto conferente con i richiami presenti

che si allontani dalle regole o dai principi generali dell'ordinamento, ma di un arbitrato che tiene conto di questi principi e di queste circostanze. Quindi, uno dei punti fondamentali sicuramente è stato

della legge 12 febbraio 1955,

coordinate e continuative. Ecco perché riteniamo che la discussione e la perimetrazione sia assolutamente corretta e riguardi l'ambito entro il quale il Presidente della Repubblica ha invitato le Camere a riflettere. l'Aula a votare in questo senso e per questa perimetrazione proposta dal relatore, senatore Castro.

Prego ciascuno di votare per sé e chiedo ai senatori Segretari di verificare.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, ricorre oggi il 34° anniversario del terremoto che colpì il Friuli. Ricordare è necessario perché il terremoto fu una vicenda dai risvolti epici, umani e religiosi, una sorta di anno zero che ha creato il modello friulano degli interventi nelle emergenze modello non facilmente esportabile perché profondamente radicato nella natura del popolo che lo ha reso possibile, ma esempio su cui fondare ogni opera di ricostruzione futura - con una classe politica che rispose compatta. È giusto continuare a ricordare, perché non c'è futuro se non c'è memoria, e un Paese non può guardare avanti se non trova le radici del suo trascorso. Fu allora una tragedia, ma da essa emerse la forza del carattere del popolo friulano, della cultura e della solidarietà. Il sisma del Friuli generò il modello della Protezione civile, che nacque lì, da quella esperienza, e lì, nella fase della ricostruzione (prima delle fabbriche e delle scuole, poi delle case ed infine delle chiese), si è prefigurato anche un modello di federalismo virtuoso, solidale, sviluppato con responsabilità dai sindaci e dalle popolazioni di ogni Comune terremotato. una lezione di buonsenso, senza litigiosità e senza conflitti.

di indicare quante persone di etnia rom salgono sul treno. Poiché a vista nessuno potrebbe o dovrebbe essere identificato per motivi etnici, ammesso che - come diceva Einstein - le etnie esistano,

del collega Pertoldi, che ha ricordato l'anniversario del terribile terremoto del Friuli. Fu un terremoto devastante, che provocò oltre 1.000 morti e 100.000 senzatetto; un terremoto che venne gestito in modo unitario da tutte le forze politiche e da tutte le istituzioni, diventando un esempio per l'Italia di come si affrontano e si gestiscono calamità di questo genere. È giusto ricordare questo anniversario, per ricordare i tanti morti, ma anche e soprattutto per ricordare come situazioni di questo genere, se affrontate con spirito unitario e costruttività, alla fine portano a grandi risultati. In sei-sette anni il Friuli venne ricostruito, 100.000 case vennero realizzate quindi un numero consistente - 100.000 vennero riparate e sistemate e venne rilanciato tutto l'apparato produttivo e culturale di quella terra.

intervengo per aggiungere alle parole importanti ed esaustive dei colleghi che mi hanno preceduto solo una notazione, non certo a margine. Quel terremoto e le dinamiche che portarono alla coscienza da parte del Paese di una serie di emergenze (in quell'occasione in particolare l'emergenza venne affrontata con particolare spirito di iniziativa e con un senso tutto italiano della solidarietà) vide al centro di quei soccorsi e anche della ricostruzione dell'alpino, che poi tutti gli italiani avrebbero continuato ancor più ad amare. Mi riferisco all'Associazione nazionale degli alpini, a tutti gli alpini friulani e a tutti gli alpini d'Italia, che in quei giorni, con grande spirito di sacrificio, misero a disposizione tutto il loro tempo, tutta la loro volontà, tutta la loro straordinaria capacità, suggellata da quella grande umanità che fa del loro il Corpo più amato dagli italiani.